Signor Presidente,

Il 14 agosto 2018, alle ore 11,13, un velivolo di EUNAVFOR Med dell'operazione Sophia

l'*Italian maritime rescue coordination center* (IMRCC) presso la Guardia costiera italiana della presenza di un barcone con circa 120 persone in navigazione con rotta Nord, a circa 40 miglia dalle coste libiche, all'interno dell'area SAR libica. Le autorità di Tripoli assumevano il coordinamento del caso, disponendo l'uscita di una propria motovedetta, che successivamente rientrava in porto a causa di un problema tecnico. Il barcone in questione continuava la navigazione in direzione nord e nella mattina del 15 agosto, esattamente alle ore 8,53, l'autorità maltese, precedentemente compulsata da quella libica con apposito messaggio, assumeva la responsabilità del caso a seguito della localizzazione, effettuata da proprie unità aereonavali, in acque SAR maltesi, in una posizione distante circa 50 miglia a sud di Malta e circa 100 miglia da Lampedusa. Durante la stessa mattinata del 15 agosto, alle ore 10,06, un aereo, sempre di EUNAVFOR Med, operazione Sophia, avvistava il barcone e nelle sue vicinanze due unità militari con numeri identificativi maltesi P52 e P61, nonché un battello ausiliario di una delle navi maltesi affiancato al barcone. La posizione da ultimo rilevata evidenziava un deciso cambiamento di rotta rispetto a quella precedentemente tenuta dal barcone verso l'isola di Lampedusa. In questo frangente, le navi militari maltesi procedevano a rifornire i migranti di viveri, acqua e giubbotti di salvataggio, come comunicato dalle autorità SAR di Malta. Alle ore 19,20 del 15 agosto anche un velivolo della Guardia costiera italiana avvistava il barcone con i migranti nell'area di responsabilità maltese che dirigeva verso Lampedusa, a circa 5 miglia dal predetto barcone. Il velivolo avvistava il pattugliatore maltese P52, che procedeva con le stesse rotta e velocità dell'imbarcazione dei migranti. Veniva altresì rilevato a una distanza di 5 miglia, ma in direzione nord rispetto al barcone, anche il secondo pattugliatore maltese P61, che risultava essere fermo. Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente indicavano la rotta ai migranti scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza SAR italiana alle primissime ore del giorno 16. Da un'analisi della situazione meteorologica e dall'esperienza maturata negli anni circa le possibilità di protrarre la navigazione con quella tipologia di imbarcazione (vale a dire stato di vetustà del mezzo, livello di galleggiabilità a bordo libero e numero di persone a bordo), constatata l'inerzia delle autorità SAR maltesi, il nostro Comando generale

per alleggerire il barcone una volta che fosse entrato nell'area di responsabilità nazionale. Per predisporsi a tale eventualità, dalle ore 20,24 del 15 agosto il Comando attuava le seguenti misure. Primo. Allertava in via preventiva le altre autorità italiane di riferimento, comunicando le proprie intenzioni e richiedendo altresì, come da prassi, al Dicastero dell'interno, qualora si fosse verificato l'ingresso in area di responsabilità SAR italiana, l'assegnazione del porto di sbarco dei naufraghi (nel gergo "*place of safety*"), secondo le procedure consolidate e concordate dal 2015 con il Ministero dell'interno, in aderenza anche all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Secondo. Sempre il Comando disponeva l'uscita in mare di due motovedette da Lampedusa (CP305 e CP324), finanziate dall'agenzia Frontex, perché partecipanti all'operazione Themis (nota missione sulla vigilanza delle frontiere europee), con l'ordine di rimanere all'interno dell'area SAR italiana, al fine di assicurare il necessario intervento solo allorquando il barcone avesse raggiunto la zona di competenza. Terzo: stante l'elevato numero dei migranti - in quel momento il numero esatto era ignoto - e la capacità di trasporto delle due motovedette GC classe 300 (massimo 110 persone ciascuna), disponeva l'avvicinamento in zona di nave Diciotti, al momento impegnata in una campagna di controllo attività di pesca a circa 20 miglia nautiche a nord-est di Lampedusa. Alle ore 00,40 il Comando generale delle Capitanerie adottava un ordine di operazioni diretto alle unità navali della Guardia costiera impegnate, che prevedeva, *in primis*, di assistere il barcone facendolo proseguire nella navigazione verso Lampedusa ovvero, in caso di criticità, l'adozione tempestiva di azioni tese ad evitare pericoli per i naufraghi, a tutela e a salvaguardia delle vite umane in mare. Già alle ore 2,49 di Lampedusa. Alle ore 00,40 il Comando generale delle Capitanerie adottava un ordine di operazioni diretto alle unità navali della Guardia costiera impegnate, che prevedeva, *in primis*, di assistere il barcone facendolo proseguire nella navigazione verso Lampedusa ovvero, in caso di criticità, l'adozione tempestiva di azioni tese ad evitare pericoli per i naufraghi, a tutela e a salvaguardia delle vite umane in mare. Già alle ore 2,49 veniva informato il Rescue Coordination Centre di Malta che il barcone si era fermato, chiedendo di adottare ogni azione finalizzata a prestare soccorso agli occupanti, dato che lo stesso si trovava all'interno dell'area di responsabilità maltese. ore 3,20 del 16 agosto, giunti a meno di quattro miglia dal limite dell'area di competenza SAR italiana, ancorché in piena zona contigua italiana, i migranti contattavano via telefono il Comando generale delle Capitanerie di porto riferendo che la situazione a bordo si era aggravata a causa del fatto che il barcone si era fermato e cominciava ad imbarcare acqua. Posto che le comunicazioni pervenute erano idonee a configurare un concreto e imminente pericolo di vita per i migranti, rafforzate dalla previsione del peggioramento delle condizioni meteo marine in zona - attenzione, c'era mare forza 4, con onde di circa 2 metri, confermato dalle unità di Guardia Costiera in area il Comando generale delle Capitanerie disponeva l'intervento immediato, alle ore 3,21, dei mezzi della Guardia costiera italiana. L'operazione di soccorso avveniva a circa 18 miglia da Lampedusa, a 70 miglia da Malta e a 97 dal porto de La Valletta. Di ciò veniva data comunicazione all'autorità maltese, che però rispondeva solo una volta intraprese le operazioni di soccorso, dichiarando oltretutto la volontà di non interferire. Tutto ciò nonostante Malta - sottolineo - fosse stata messa a conoscenza, per iscritto, che il barcone era in procinto di affondare con i propri occupanti. Con lo stesso messaggio si chiedeva il contestuale porto di sbarco dei migranti a Malta. Le unità maltesi, già precedentemente individuate in navigazione nei pressi del barcone, si erano nel frattempo allontanate una volta giunte in prossimità dell'area di responsabilità SAR italiana. Al momento del soccorso le unità più vicine e utilmente impiegabili risultavano, pertanto, le sole motovedette della Guardia costiera italiana. Concluse le operazioni, al fine di verificare l'eventuale presenza di altre persone a bordo, l'equipaggio della motovedetta CP-324 effettuava una ricognizione del barcone, constatando un elevato livello di acqua nel locale motore. Attesa la pericolosità e le critiche condizioni di stabilità del mezzo, i militari lasciavano immediatamente l'imbarcazione, dopo aver accertato che non vi erano altre persone a bordo. A causa dell'elevato numero di persone soccorse, che a fine operazione risulteranno essere 190, per il peggioramento delle condizioni meteorologiche e l'impossibilità di utilizzare l'*hotspot* di Lampedusa, i naufraghi venivano suddivisi tra le due motovedette intervenute e successivamente trasferiti sulla nave Diciotti, nel frattempo avvicinatasi in zona, sulla quale erano imbarcati un *team* sanitario e mediatori culturali in grado di fornire assistenza. Nelle ore seguenti, sulla base del *triage* sanitario effettuato a bordo dal personale medico imbarcato, veniva effettuata l'evacuazione medica a favore di 13 migranti su Lampedusa: sette infermi e sei accompagnatori. Alle prime luci del giorno 16, il Comando generale delle Capitanerie disponeva un sorvolo di un velivolo della Guardia costiera, già impegnato in attività di sorveglianza marittima, per una ricognizione della zona, rilevando l'assenza del barcone, ma riscontrando chiare tracce di un affondamento, quali iridescenze da idrocarburi, diversi giubbotti di salvataggio sparsi in acqua ed elementi strutturali di un'imbarcazione riconducibile al barcone in parola. Questi ultimi elementi ci inducono a concludere che, senza l'intervento concreto e diretto della nostra Guardia costiera, molte di queste persone sarebbero senz'altro morte. Nel frattempo, la nave Diciotti con i rimanenti 177 migranti a bordo, nelle more dell'individuazione del *place of safety*, rimaneva nelle vicinanze di Lampedusa sino al 19 agosto. In attesa della definizione con le autorità maltesi delle operazioni di sbarco, che ad avviso delle autorità italiane permaneva in capo alla responsabilità di quel Paese, la nave Diciotti effettuava nella tarda sera del 20 agosto scalo tecnico nel porto di Catania, su indicazione dei vertici del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, in attesa dell'eventuale indicazione del *place of safety* da parte anche del Ministero dell'interno. Il giorno 22 agosto, non appena avuto cognizione della loro presenza a bordo, con l'unità in porto a Catania, il Dicastero dell'interno autorizzava un primo sbarco dei 27 minori non accompagnati nei centri di accoglienza dedicati della provincia di Catania, anche in conseguenza delle interlocuzioni con il procuratore della Repubblica dei minorenni di Catania. Sin dai giorni successivi all'arrivo nel porto di Catania, esperiti inutilmente i tentativi di intesa con le autorità maltesi, che confermavano la loro posizione di non voler interferire e di non assumersi alcuna responsabilità *(**Commenti avviava interlocuzioni con le istituzioni europee, al fine di condividere un piano di ripartizione dei migranti, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dello sbarco verificatosi nel porto di Pozzallo, nello scorso mese di luglio. Il 24 agosto veniva convocata a Bruxelles una riunione, alla quale ovviamente partecipavano anche i delegati del Governo italiano,

di Catania. L'operazione è stata conclusa senza alcuna criticità nella notte tra il 25 e il 26, con il loro trasferimento presso l'*hotspot* di Messina. Tutti i migranti, al momento dello sbarco, hanno manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale. terminato il dettagliato resoconto, formulo qualche osservazione e considerazione insieme. Le operazioni sopra descritte hanno inteso sempre privilegiare la salvaguardia delle vite umane e della dignità delle persone… …coniugando tale intendimento con l'altrettanto necessario rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa internazionale e convenzionale sul salvataggio in mare e sul diritto d'asilo dei migranti. Le autorità maltesi, pur avendo assunto formalmente sin dall'inizio la responsabilità del coordinamento dell'intervento, con il trascorrere delle ore hanno dimostrato - e attestato concretamente - l'intendimento di non procedere alle operazioni di soccorso, limitandosi a indicare ai migranti, anche scortandoli, la rotta nella direzione dell'area SAR di competenza italiana. Si è continuato a chiedere a Malta, senza ottenere alcuna risposta, di indicare il porto di sbarco. Infatti, nonostante la situazione di grave pericolo per le persone - evidenziata dallo stato di precarietà del barcone, inabissatosi poi nelle ore successive

Va comunque precisato che, nei giorni in cui la nave Diciotti è stata ormeggiata nel porto etneo, è stata costantemente assicurata ogni necessaria assistenza ai migranti. Non è stata, invece, una bella pagina per l'Europa, che ha perso l'occasione per dare concretezza e attuazione immediata a quei princìpi di solidarietà e responsabilità che pure vengono costantemente e diffusamente evocati, a destra e a manca, come valori fondativi dell'intero ordinamento eurounitario. Il Governo italiano ha ribadito, fin dall'avvio del caso Diciotti, la propria convinzione che esso dovesse necessariamente essere affrontato in linea con i princìpi di solidarietà e di condivisione tra i Paesi dell'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori. Si è tentato dapprima, come ho già detto, di chiamare alla responsabilità le autorità maltesi, e si è comunque lavorato assiduamente affinché si realizzasse una ripartizione delle persone soccorse in mare; ripartizione che, peraltro, non era affatto utopistica, dal momento che era avvenuta nei casi di emergenze anche in settimane precedenti. Ricordo la nave Lifeline, con a bordo 234 persone, sbarcate a La Valletta nel giugno scorso. Ricordo la nave Open Arms, con a bordo 60 persone, sbarcate a Barcellona nel luglio scorso. Ricordo anche da noi il barcone con a bordo 450 persone, sbarcate a Pozzallo nel luglio scorso. Ancora, un'altra volta, la Open Arms, con a bordo 87 persone, sbarcate ad Algeciras ad agosto. Infine, l'Aquarius, con 141 perone a bordo, sbarcate a La Valletta ad agosto. Già prima, quindi, che si verificasse il caso Diciotti, e ancora successivamente ad esso, il Governo italiano si è fatto promotore di una insistita e determinata iniziativa, volta a sollecitare le istituzione europee affinché vengano tempestivamente attuate le conclusioni adottate, all'unanimità, all'esito del Consiglio europeo dello scorso fine giugno. Il Governo italiano sta ribadendo agli altri Stati membri dell'Unione europea e alle istituzioni europee la ferma convinzione che sia improcrastinabile l'avvio della definizione di un meccanismo stabile e sostenibile per la gestione complessiva delle fasi di sbarco, redistribuzione e rimpatrio. Stiamo registrando segnali di avvicinamento nel segno di una comune, speriamo sempre maggiore, consapevolezza degli Stati membri che se non si lavorasse ad un simile meccanismo non solo non si darebbe coerente attuazione alle decisioni prese dall'ultimo Consiglio europeo, ma si verrebbe meno all'impegno, alla solidarietà e all'equa ripartizione di responsabilità che sono specificamente previsti dagli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La nostra politica sull'immigrazione non risponde a logiche emergenziali o a contingenze transeunti. Abbiamo fatto di più: abbiamo proposto un'articolata e complessa strategia che mira ad offrire una regolamentazione e una gestione dei flussi migratori in via strutturale, consegnata ad un documento che abbiamo proposto alle istituzioni europee sin dai primi incontri sul tema, articolato in sei premesse e dieci obiettivi. Tale proposta è quindi documentata anche nelle nostre posizioni ufficiali che abbiamo successivamente sostenuto in occasione dei vari consessi europei. È una politica che muove, fin dalle prime affermazioni, dal riconoscimento della tutela dei diritti fondamentali di tutti coloro che hanno diritto all'asilo e alla protezione umanitaria e mira ad adottare iniziative di tutela di questi migranti sin dai Paesi di origine e anche nei Paesi di transito. Quello che è cambiato, rispetto al passato, è che l'Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo, anche solo involontariamente, a incrementare ed incitare il traffico di esseri umani e supplendo alla responsabilità che spetta all'Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro. Grazie per la vostra preziosa attenzione.

credo che questa, come altre, non sia stata una pagina gloriosa, né per il nostro Paese, né per gli Stati membri dell'Unione europea. Questo è il fallimento dell'Europa sovranista, dell'Europa degli Stati che sempre, però, viene confusa con l'Europa comunitaria (è bene che ci chiariamo anche nel vocabolario) e io credo che andare avanti sulla rivendicazione delle sovranità nazionali, salvo quando ci fa comodo, non sia una buona politica.

o, come diceva Pannella, l'Europa delle patrie, ci porta solo a degli scontri di cui, di tanto in tanto siamo i perdenti. Quello che serve nella costruzione della patria europea che si aggiunge, ovviamente, all'appartenenza nazionale di ciascuno di noi come valore aggiunto: questo è l'obiettivo cui dobbiamo mirare. Quindi basta con i *summit* e con l'assunzione "su base volontaria" (viene da ridere, francamente, se non da piangere) delle conclusioni dei vertici di volta in volta. plauso va alla Guardia costiera italiana, ma rimane il fatto - e lo ripeto ancora - che questa non è stata una bella pagina, né per gli Stati membri dell'Unione europea, né per il nostro Paese, né dal punto di vista politico, né da quello diplomatico; e non parliamo delle procedure, tantomeno nelle fasi successive.

di portare avanti il progetto europeo e di non essere così permalosi. Se per caso un'agenzia delle Nazioni Unite, che ha già fatto una missione nel 2016 in Italia, senza che nessuno si scandalizzasse, ma anzi con grande cooperazione del Governo, del Governo, annuncia un'ispezione nel nostro Paese, non è il caso di minacciare subito di togliere i fondi. Non è così - a mio avviso - che si conquista la credibilità nell'ambito internazionale. Non è una gara a chi la spara più forte.

*(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente del Consiglio, su quella nave c'erano soprattutto cittadini dell'Eritrea, un Paese dal quale si fugge per via di un servizio di leva a tempo indeterminato, sotto le armi o nelle tante forme di lavoro del cosiddetto servizio nazionale, che è un modo che si è dato il regime per mantenere il controllo sull'intera società, con oppositori *leader* religiosi e obiettori di coscienza che restano in carcere in attesa di un processo e dell'entrata in vigore di una Costituzione che definisca diritti e doveri dei cittadini. Si scappa da quella vecchia colonia italiana e da tante altre parti dell'Africa perché si è spinti dalla disperazione e ci si vuole liberare da condizioni di oppressione, di fame e persecuzione. Le donne e gli uomini della Diciotti portavano tutti i segni di violenza subita nel corso del loro viaggio per raggiungere le coste libiche. Il capitano ha detto ad alcuni deputati che non sapeva bene come comportarsi dopo aver letto un messaggio su Facebook del Ministro dell'interno che entrava in contraddizione con gli ordini che aveva ricevuto. Insomma, si era creata una situazione assurda e paradossale. Il fatto che Malta abbia sbagliato non giustifica la gestione italiana. A noi questo modo di intendere la diplomazia internazionale ed europea non convince, anche perché è poco efficiente, e non sono io a dirlo. Dinanzi a quanto accaduto in questi mesi, da parte dell'Europa non c'è stata una sola apertura nei confronti delle ragioni italiane, semmai un passo indietro con la ricollocazione non più obbligatoria dei richiedenti asilo tra i Paesi europei. È la riprova che l'Italia, se deciderà di andare a braccetto con i Paesi del Gruppo di Visegrád, non vedrà mai riconosciute le sue ragioni. È chiaro che l'Europa deve fare la sua parte, soprattutto se l'instabilità libica dovesse degenerare e dovessero ricominciare con forza le partenze, ma da più di un anno l'emergenza è finita, gli sbarchi sono diminuiti del 80 tanto che a inizio estate si contavano più arrivi in Spagna che nel nostro Paese. Adesso dobbiamo avere a cuore la stabilità della Libia e su questo, nelle scorse settimane, abbiamo ascoltato parole condivisibili e di buon senso da parte di tutto il Governo.

la frequentazione di corsi di integrazione e il rispetto dell'obbligo scolastico. Per questo, signor Presidente del Consiglio, ci aspettiamo su siffatto tema un cambio di passo. non gesti eclatanti, ma un'opera paziente e costante di responsabilizzazione dell'Europa e un lavoro sull'Africa e per l'Africa. A noi questo modo di fare non piace e siamo convinti non piaccia neppure a lei, signor Presidente del Consiglio, che si è sempre distinto per rispetto del suo ruolo e delle istituzioni. Le chiediamo, quindi, di correggere la rotta del suo Governo e di alcuni suoi Ministri.

l'Italia è uno Stato di diritto. E lei, presidente Conte, da uomo di legge e come Presidente del Consiglio, dovrebbe saperlo e ricordarlo ai suoi colleghi di Governo. Nei lunghi giorni in cui si è consumato il caso della nave Diciotti, la sua voce non si è sentita, se non per ribadire sempre un solo concetto: «Condivido quanto sta facendo il ministro Salvini»; salvo poi lasciar trapelare le perplessità attraverso spifferi e retroscena. questo non la solleva dalle responsabilità, anzi evidenzia la sua debolezza: lei, signor Presidente, è in balia dei suoi dante causa - per usare un termine a lei ben noto come civilista - e della lotta all'ultimo sondaggio che corre tra Lega e Movimento 5 Stelle; è relegato al ruolo di vaso di terracotta tra vasi di ferro. Avremmo voluto sentirle dire ben altro. Avremmo voluto vederla difendere strenuamente l'onore dell'Italia, delle sue leggi, della sua storia e delle sue istituzioni. Ciò che avete fatto non è servito proprio a nulla. A ben guardare, la prova muscolare del Ministro dell'interno, proprio a partire dai rapporti con i vostri alleati in Europa, non ha sortito alcun effetto, Non ci risulta che i Paesi del Gruppo di Visegrád - a partire dal premier Orbán, con i quali sperate non di cambiare nel profondo, ma di distruggere l'Europa unita

Questi comportamenti hanno smentito platealmente l'accordo su base volontaria per il quale lei stesso esultava a fine giugno dopo il Consiglio europeo. Lei ha permesso che le ragioni della propaganda leghista prevalessero sugli accordi internazionali, sulla dignità e sull'onore del nostro Paese. Forse oggi si sarebbe dovuto presentare il ministro Salvini al posto suo, ma è toccato a lei quest'ingrato compito. Ancora una volta, avete fatto i forti con i deboli, tenendo in ostaggio - è questa la parola giusta 177 uomini, donne e bambini, vittime nei campi libici di torture indicibili e stupri, umiliando loro, come esseri umani, la loro storia e la nostra. persone che, vista la loro nazionalità, hanno ogni diritto, in base all'articolo 10 della nostra Costituzione, di chiedere asilo politico nel nostro Paese, sin da quando si trovano sul territorio italiano, su una nave come quella della Guardia costiera. Il fatto che oggi stiano cercando di andarsene altrove in Europa non modifica di una virgola le colpe di questo Governo. Presidente Conte, lei ha permesso al suo Ministero dell'interno di delegittimare in diretta Facebook un altro potere dello Stato, il cui unico errore è stato quello di fare il proprio lavoro, come prescrive la Costituzione e come prevedono quelle leggi che il Parlamento ha approvato. Ma io le chiedo: non ha sentito il dovere di alzare il telefono e spiegare al ministro Salvini che nessun voto popolare mette un politico al di sopra della legge? [**Presidenza del vice presidente cosa significa che il suo Governo e i suoi membri possono scegliere di porsi al di sopra della legge, per perseguire le proprie idee e azioni politiche? Lei, signor Presidente, sottoscrive queste parole? Voglio dire ai miei ex colleghi che svolgono la funzione affidata loro dalla Costituzione che sono e sarò loro vicino e so che mai si faranno fermare o intimidire da simili atteggiamenti. Avete ottenuto il risultato di cacciare le navi delle ONG dal mare, ma - come abbiamo scoperto - i naufragi e le morti continuano. Non avete risolto alcun problema. State solo cercando di impedire che questi eventi si conoscano. Il vostro impegno dovrebbe essere salvare vite umane e affrontare le dinamiche migratorie con lungimiranza, perché la storia non vi assolverà: non basterà appellarsi all'egoismo altrui. Del resto, in questi cento giorni non c'è un solo atto, un solo risultato apprezzabile da parte del Governo Lega-Cinque Stelle, se non un braccio di ferro miseramente perso; e rimane una manciata di *tweet* e di *post* Lo dica al ministro Salvini: continueremo a contrastare la sua politica basata sulla paura, sulla discriminazione e sulla propaganda a spese dei più deboli. La La contrasteremo in questa Aula e la contrasteremo nel Paese, come hanno dimostrato le manifestazioni a Catania e a Milano. Diciamocelo francamente: come avvocato dei cittadini non sta facendo una bella figura. C'è forse da augurarsi che ella sostenga presto l'esame per trasferire la sua cattedra a Roma. *(Applausi dai la cordialità personale nei suoi confronti, non vediamo l'ora che torni a fare il mestiere che meglio le riesce e si possa, ancor prima, archiviare la stagione di questo Governo della paura, Governo della paura! *(Applausi

voglio innanzitutto chiarire la piena e totale solidarietà di Fratelli d'Italia al Ministro dell'interno per la follia di ritrovarsi indagato per sequestro di persona quando, invece, si è limitato a fare il proprio dovere. A prescindere da ciò che vorrebbe qualcuno in quest'Aula, in Italia è ancora non consentito entrare illegalmente. È compito del Ministro dell'interno impedire che si possano verificare fenomeni di immigrazione illegale sul territorio italiano. Il Ministro dell'interno ha fatto il suo dovere e non ha senso che sia oggi indagato. Piuttosto, appare bizzarro che negli ultimi anni nessuno abbia mai immaginato di indagare i precedenti Governi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per danno erariale.

li accogliamo e li manteniamo a spese degli italiani. Ma dopo il primo anno, quando i dati ufficiali del Viminale ci dicono che solo il 15 per cento di chi sbarca in Italia ha diritto alla protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra o secondo la protezione sussidiaria dell'Unione europea, allora no, non si può per altri cinque anni far finta di nulla e continuare a far entrare persone e mantenerle sul nostro territorio. Lì sì ci sarebbe materia per indagare per favoreggiamento dell'immigrazione illegale e danno erariale. Vediamo se qualcuno intenderà farlo con la stessa fermezza.

Gli immigrati della nave Diciotti non sarebbero dovuti arrivare sul territorio italiano. Il problema non è dove far sbarcare gli immigrati (in Italia, a Malta o in un altro porto) né, se poi li facciamo entrare in Italia, dove distribuirli. Non è questa la strada. Lungi da me difendere Malta, ma sappiamo tutti che Malta ha meno di 500.000 abitanti e che è il Paese dell'Unione europea con la più alta densità di popolazione. non possiamo immaginare che una popolazione di 500.000 abitanti accolga i 500.000 clandestini sbarcati in Italia, perché ciò vorrebbe dire segnare la fine di Malta. Non è questa la strada. Malta difende la propria sopravvivenza, cosa che dovremmo fare anche noi e cosa che dovrebbe fare l'Europa. Abbiamo più volte sentito dire che l'Africa in Italia non ci sta. È vero. Vi comunico che neanche in Europa ci sta, perché l'Africa ha un miliardo e 200 milioni di abitanti, molti dei quali avrebbero legittimamente l'ambizione di venire a vivere in Europa. Non possiamo allora immaginare che la soluzione sia di non far sbarcare la gente solo in Italia, ma distribuirla in Europa e, quindi, far invadere non solo l'Italia, ma l'intera Europa. È questa la strategia del Governo? Capiamoci. La soluzione di chi si dichiara sovranista è un'altra: difendere i confini esterni dell'Unione europea, come fanno i popoli dell'Est Europa, come fa tutta l'Europa, come fa la Spagna e come, purtroppo, non l'ha fatto l'Italia in questi anni. Come si difendono i confini esterni dell'Unione europea? Si difendono con un blocco navale a largo delle coste libiche, per impedire ai barconi di partire. Abbiamo sentito il ministro Trenta dire che il blocco navale non si può fare, perché è un atto ostile. Eravamo abituati a sentire speravamo che cambiassero. E, quindi, diremo alcune cose. C'è una misura che l'Italia, con il sostegno dell'Unione europea, potrebbe attuare subito: presidiare il mare davanti alla Libia, e l'ONU appoggerebbe questa iniziativa. E lo dice non un pericoloso sovranista, ma Bernardino León, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia. Ma ancora: Unione europea, blocco navale in Libia contro le morti in mare. Queste sono le conclusioni del vertice informale di Malta del 3 febbraio 2017; il titolo è quello de "l'Unità" e non della "Voce del Patriota".

che è l'ultimo *Premier* italiano ad aver fatto un blocco navale, nel 1997, per impedire ai barconi che partivano dall'Albania di arrivare in Italia, schierando la nostra Marina militare per fare quello per cui è nata. Abbiamo una Marina militare

si riferiscono all'occasionale salvataggio in mare di una nave in difficoltà. Tutte quelle norme si riferiscono al caso di un peschereccio che, mentre sta facendo tutt'altro, si imbatte in una nave in difficoltà e quindi ha il dovere di soccorrere chi sta affogando, così come lo Stato più vicino ha il dovere di accogliere il peschereccio con a bordo i naufraghi. Questo è il salvataggio in mare. Non esiste alcuna norma di diritto internazionale che prevede

o la Libia controlla i propri confini e le proprie coste, e allora la partenza dei barconi è un atto ostile che giustifica il blocco navale italiano; oppure non controlla le proprie coste, e allora il blocco navale non è un atto ostile contro la Libia. Questo è il diritto internazionale. Il diritto internazionale dice che l'unica azione che oggi l'Italia può porre in essere per difendere la legalità è il blocco navale e non impedire ai disperati di sbarcare in Italia,

nel territorio dell'Unione europea coloro che vengono salvati, a norma del diritto internazionale, dovrebbero essere trasferiti in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri; qui un trattamento rapido e sicuro consentirebbe, con il pieno sostegno dell'Unione europea, di distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà. Perché il Governo italiano non ha ancora istituito i centri sorvegliati dove, per quanto deciso dal Consiglio europeo del 28-29 giugno, devono essere portati coloro che entrano illegalmente in Italia?

La Merkel, paladina dell'integrazione europea e delle anime belle della Unione europea, ha di recente istituito tali centri chiamandoli «centri di ancoraggio».

Signor Presidente del Consiglio, la ringraziamo di essere qui oggi a riferire sul caso della nave Diciotti. La ringraziamo di avere fatto sentire oggi la sua voce, quella che - a nostro giudizio - avrebbe dovuto far sentire forte e chiara nelle nove giornate in cui abbiamo assistito al perpetrarsi di un sopruso nei confronti non solo dei migranti, in spregio alle regole internazionali e nazionali, ma anche dei principi che regolano il funzionamento del nostro Stato nei rapporti tra i corpi dello Stato stesso. Tornerò su questo, ma mi permetta di fare un breve *excursus* sugli accadimenti precedenti. Lei, il 29 giugno, dopo il vertice dei Capi di Stato europei, ha dichiarato con enfasi che ha lottato fino alla fine e che l'Italia ha rivoluzionato il tavolo. ha detto al Paese che finalmente l'Italia ha saputo affermarsi e da quel giorno non era più sola. Noi siamo rimasti un po' perplessi perché dalla lettura del documento finale del vertice abbiamo scoperto che i ricollocamenti, prima obbligatori, non rispettati da tutti

Ma tant'è. Avremmo voluto crederle, perché non c'è dubbio che l'Europa in questi anni si è spesso voltata dall'altra parte su un problema, come quello della crisi dei flussi migratori dopo le tensioni e instabilità nel Nord Africa e la guerra in Siria, che non può essere considerato italiano. Sappiamo che chi scappa cerca di arrivare in Europa con i barconi, non in Italia, e su questo siamo d'accordo, signor Presidente. Però abbiamo pensato che quella trasformazione da obbligatoria a volontaria non fosse una buona nuova per il nostro Paese, nonostante la sua enfasi. Ma ripercorriamo le vicende delle navi con carico di dolore e di sofferenza e della chiusura dei porti. All'inizio di giugno c'è il primo braccio di ferro tra il Ministro dell'interno e la nave Aquarius che ha salvato i migranti: la (ONG) e il Ministro sostiene che non possono sbarcare in un porto italiano. La crisi si risolve con la disponibilità della Spagna e di altri Paesi europei ad accoglierli: già i primi migranti sono stati presi in ostaggio senza che vi fosse emergenza. Poi è la volta della nave Samuel Beckett della Marina irlandese, che fa parte della missione europea EUNAVFOR Med, di cui l'Italia ha il comando con l'ammiraglio Credendino. Sulla base delle regole della missione, i migranti salvati devono essere sbarcati nel primo porto sicuro, ma il Ministero dell'interno blocca lo sbarco. Immagino lo stupore degli irlandesi e anche degli altri Paesi: un ordine di un ammiraglio italiano (a capo di una missione europea, ma è un ammiraglio italiano) fermato dal blocco di un Ministro dello stesso Paese. Dopo un po' di traccheggiamenti i migranti vengono fatti sbarcare. Il Ministro dell'interno in quel caso dichiara che a Innsbruck, nella riunione dei Ministri dell'interno, avrebbero modificato le regole di EUNAVFOR La Difesa rappresenta che non è un compito di sua competenza; infatti, se ne parlerà a Vienna alla fine di agosto tra alcuni Ministri della difesa e degli esteri nella sede competente, ma la missione Sophia viene confermata con le regole precedenti. L'Italia non si sfila - secondo me giustamente - perché quella missione al centro del Mediterraneo è fondamentale per i nostri interessi strategici, compreso il contenimento dei flussi. Tuttavia, le precedenti roboanti dichiarazioni, che hanno funzionato mediaticamente, avrebbero fatto pensare a un'azione diversa e, se da un lato ritengo positivo che l'Italia sia rimasta, questo però fa perdere credibilità all'Italia in Europa. Non crede, signor Presidente del Consiglio, che la reputazione e il posizionamento dell'Italia rispetto agli alleati chiamino in causa anche lei? Arriviamo così al caso della nave

signor Presidente del Consiglio, le unità militari italiane avevano ancora il permesso di attraccare nei porti italiani, ad agosto no. Dalla notte fra il 15 e il 16 agosto e la notte fra il 25 e il 26 agosto in Italia viene sospeso il diritto. La nave Diciotti rimane vicina a Lampedusa dal 16 agosto mattina fino al 19 e arriva a Catania il 22, ma i migranti possono sbarcare solo nella notte tra il 25 e il 26 agosto: sette giorni in mare e quattro in porto su una unità militare italiana, con bambini, persone malate e donne. Peraltro, quell'unità militare è già suolo italiano, signor Presidente del Consiglio, e di fatto è stato trattato un Corpo militare dello Stato (la Guardia costiera) come una nave straniera. Non c'era alcuna motivazione, né di emergenza né di ordine di sicurezza pubblica, per creare questa situazione. I migranti erano già stati salvati da una nave della Guardia costiera, non da una ONG che voi avete messo al bando, la Guardia costiera è un Corpo militare dello Stato con compiti di ricerca e salvataggio in mare e ripeto che tale nave è già territorio italiano. Si crea quindi ad arte un conflitto fra Corpi dello Stato: il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli non dice nulla, ma neppure lei dice nulla in tutto questo tempo, lei che è il Presidente del Consiglio e che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

per tutti quei giorni quella nave non ha potuto attraccare in porto. Lei questo ci doveva spiegare questa mattina. La Guardia costiera italiana interviene a 17 miglia da Lampedusa - ce l'ha detto anche lei questa mattina, signor Presidente

molti sono in Italia, come vediamo anche dagli spostamenti che stanno facendo all'interno del nostro Stato. E ora non interessano più: interessavano solo quando erano su quella nave. Quindi, il problema era non l'accoglienza in Italia, perché oggi sono qui, ma avere degli ostaggi per una trattativa diplomatica con l'Europa. Signor Presidente del Consiglio, una Nazione degna di questo nome non si comporta così. Lei ha detto che non è stata una bella pagina per l'Europa. Credo anche io che l'Europa abbia sbagliato a voltarsi dall'altra parte, ma non è stata una bella pagina neppure per l'Italia. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha giurato su una formula molto simile a quella su cui giurano i militari. I militari giurano seguente modo: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni». Lei, però, ha messo quegli uomini e quelle donne che così hanno giurato in un grave disagio, non salvaguardando le loro funzioni. Le leggi e la Costituzione vengono prima della volontà di qualsiasi Ministro, chiunque esso sia. Spero si renda conto di quanto grave e destrutturante sia stata la sua assenza; una pessima figura per l'Italia, in barba al diritto internazionale, alle leggi, agli obblighi italiani e ai più elementari principi di umanità.

Non crediamo più a queste mistificazioni della realtà, perché sul tema dell'immigrazione il Governo si è mosso fin da subito in modo giusto

Mi sembra che la maggioranza abbia condiviso il fatto che l'importante è salvare vite umane, che è il primo aspetto fondamentale; dopodiché si tratta di impostare una strategia e una politica per cercare di cambiare davvero l'Europa ed è quello che è stato fatto, perché comunque dei risultati ci sono. Qualcuno può non vederli e far finta che non ci siano, ma questa politica ha prodotto un risultato efficace: oggi gli immigrati non possono più sperare di prendere un barcone e arrivare in Italia come se nulla fosse. In effetti, rispetto al passato, oggi è più difficile arrivare in Italia e gli sbarchi sono diminuiti.

giugno e luglio del 2018 ne sono sbarcate solo 5.080, quindi 30.000 in meno. Ripeto, quindi, che i risultati si vedono, sono chiari e non si possono negare. Tra l'altro, la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato che è dimezzato il numero dei morti, a testimonianza del fatto che il vero gesto umanitario è fermare gli sbarchi: incoraggiare l'esodo significa aumentare il numero di morti nel Mediterraneo e condannare la gran parte di quelli che arrivano un futuro di fame, schiavitù e delinquenza. poi dato un segnale forte all'Unione: con questa vicenda sono emerse le vere contraddizioni di molti Paesi europei che, se a parole fanno i campioni dell'accoglienza, nei fatti non accettano poi la redistribuzione. È vero, infatti, che si può discutere sulla redistribuzione obbligatoria o volontaria, ma, anche quando era obbligatoria,

Additare quindi l'Italia come cattivo esempio di accoglienza, salvo poi voltarsi dall'altra parte a Ventimiglia o a La Valletta, è assolutamente assurdo. Se il messaggio è che ognuno faccia da sé, a questo punto è giusto che l'Italia si muova di conseguenza, per cui avanti così, signor Presidente del Consiglio. Avanti così con il Governo.

Stando alle dichiarazioni virgolettate del comandante della nave risulta che: «Non c'era emergenza sanitaria», «La situazione era più che soddisfacente», «I migranti mangiano e stanno bene e non hanno la sensazione di essere sequestrati». Per di più, una volta sbarcati, da tanto che erano affamati, ben 75 su 143 rifiutano vitto e alloggio e si dileguano, con la conferma che quella degli scheletrini che scappano dalla guerra è una farsa.

ovviamente per tentare di impietosire i cittadini, che una successiva verifica ha dimostrato essere immagini del 2011 e del 2014 che non riguardano assolutamente fatti accaduti in Libia. Purtroppo questo è quello che sta succedendo. Come vedete, le panzane del politicamente corretto ormai sono state svelate e la gente non crede più a queste mistificazioni della realtà. Lo ripetiamo: la verità è che non basta farli arrivare qui da noi e poi e poi voltarsi dall'altra parte, lasciandoli girovagare nelle stazioni, nei giardini pubblici, in preda alla criminalità organizzata, senza dare loro una vera prospettiva di vita. Meglio bloccare i flussi, come sta facendo il Governo, e lavorare affinché nasca un'Europa che crei porti sicuri in Libia e centri di identificazione in Africa, per fare in modo che arrivino qui i veri profughi, le persone che davvero scappano dalla guerra e hanno bisogno del nostro sostegno.

Quindi, per concludere, siamo soddisfatti della politica, bisogna andare avanti con coraggio, con determinazione e coerenza, che sono le cose che alla fine ci chiede la gente, anche perché la gente stessa, il popolo, i cittadini dicono che quando si è nel giusto bisogna andare avanti: *vox populi, vox Dei*.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, la ringraziamo per la ricostruzione puntuale dei fatti, degli orari e delle date, tuttavia, come vedrà, l'aspetto politico generale lascia molto perplesso il Gruppo di Forza Italia. Condividiamo una politica di maggiore fermezza sul fronte dell'immigrazione, che fa parte delle politiche che abbiamo attuato quando abbiamo avuto ruoli di Governo e delle proposte con le quali ci siamo presentati alle elezioni. Abbiamo ritenuto, colleghi del Partito Democratico, un errore

sulle organizzazioni non governative, qualche collega residuo della precedente legislatura lo ricorderà, che determinò un'inversione di tendenza rispetto alle scorribande eccessive delle ONG.

Presidente Grasso, ho letto però questa mattina sui giornali che il procuratore della Repubblica di Genova, pur avendo inchieste molto più urgenti da fare, rilascia un'intervista al giorno per spiegare alla Lega come deve pagare e saldare i debiti e altre cose. Parlo di Genova per non parlare di Agrigento per ragioni che potrebbero investire la nostra Giunta. Il procuratore Cozzi da fare ne ha, presidente Grasso. Lei che ha fatto riferimento a suoi ex colleghi, gli faccia una telefonata; mi pare che a Genova cose da indagare ce ne siano; ogni giorno un consiglio, un'istruzione: si paga così, comprare i lingotti, fate quest'altro... Sembra un consulente finanziario, non un procuratore della Repubblica italiana.

dal Gruppo FI-BP)*: alcuni votano come noi, ritenendo ingiusta quell'accusa; altri, invece, stanno lì pronti col palo e la forca. Si dirà: pensiamo all'Italia e non all'Ungheria, ma tutto si tiene. Le voglio anche ricordare che ci sarà un vertice straordinario dell'Unione europea nei prossimi giorni nuovamente sull'immigrazione. Prenda esempio dal vice presidente del nostro partito, presidente del Parlamento europeo Tajani, che ha intimato ieri a Junker di andare con proposte concrete di azione contro l'immigrazione clandestina, e non fare questi vertici inutili,

non avesse capito che cosa le dicevano gli altri *partner* europei che le hanno voltato la faccia nel mese di agosto! Non c'era quell'accordo. Scherzo e mi scusi: problemi di traduzione o problemi politici? A mio avviso, problemi politici perché sono certo che lei l'inglese lo conosce moltissimo, di sicuro più di me. Credo che noi dobbiamo dare un'agenda e dei consigli al Governo; è vero, non bisogna intervenire in Libia (il Ministro della difesa è andato via); gli scarponi sul terreno, vecchia questione delicata. Noi stessi dicemmo che la guerra in Libia nel 2011 era un errore, ma dire che nessuno interverrà incoraggia le milizie, gli scontri. *(Applausi dal Gruppo finale per evitare una guerra civile e una fuga scomposta. Le ricordo - altro che nave Diciotti! - che ci sono almeno 10.000 terroristi tra quelli che in Libia sono pronti a partire verso l'Italia. Oggi è il 12 settembre, non è l'11, sono passati alcuni anni, ma i problemi del terrorismo fondamentalista ancora agitano l'Europa. Le dico allora rapidamente, Presidente,

Quindi, la Guardia costiera che dipende dal Ministero delle infrastrutture è un problema che ponemmo anche in Parlamento: va chiarito chi deve dare le direttive di fronte a fenomeni di questo tipo. La Solidarietà europea, le ho già detto, non c'è stata, nonostante i suoi annunci trionfali a fine giugno. C'è l'occasione del prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo; si faccia valere con sottotitoli, traduzioni simultanee e quello che vuole. lei ha detto, consigliato dalla sua dottrina giuridica e dai consiglieri diplomatici, che Malta non ha voluto interferire. Presidente, Malta se n'è fregata del destino di questi sventurati, in questa e in altre occasioni!

con il linguaggio diplomatico che si deve a un Presidente del Consiglio, ha evidenziato la viltà di Malta. C'è la SAR di Malta; quell'area di controllo dà alla stessa Malta dei benefici di varia natura economica. Ebbene, non si possono avere i benefici e poi scaricare sugli altri tutte le disgrazie del mondo! *(Applausi dal Gruppo*

quando non c'erano i trafficanti di clandestini che simulavano o creavano le tragedie marine per essere trasportati da altri Paesi. Apra un tavolo per rivedere la Convenzione del mare da cui dipende l'azione della Guardia costiera, i soccorsi dovuti e non dovuti.

è servita a trasportare clandestini. Avete chiesto che gli sbarchi di quella missione non fossero solo in Italia. Vi hanno risposto di no perché non contate nulla a livello internazionale e quindi vi dicono «stiamo tutti

ha dovuto citare in audizione il Trattato di amicizia italo-libico del 2008: chi era il Presidente del Consiglio che ha fatto la politica dell'amicizia, del blocco delle partenze e degli investimenti in Africa? Faccia un esame in italiano e risponda correttamente, non le darò consigli. Infine, per quanto riguarda la situazione della Libia, un intervento è giusto: ci sono terroristi, c'è un disastro. Anche oggi leggevo un'intervista dell'ineffabile rappresentante Quello precedente, Bernardino León, ad un certo punto ha lasciato l'incarico all'ONU e si è fatto assumere da un fondo sovrano di un Paese arabo perché veniva pagato di più. Ora c'è un altro rappresentante dell'ONU che non so cosa farà da grande ma che oggi in un'intervista si è si possano fare le elezioni a dicembre in Libia. Noi vorremmo che in tutto il mondo si votasse sempre, ma dove li fanno i seggi? Nei *bunker*, con le sparatorie? Come si vota, con un tiro a segno? L'ONU sia realista e invece di dare lezioni all'Italia sul razzismo che non c'è,

Lei l'esame di inglese lo avrebbe superato, il suo Governo l'esame di qualità non lo supererà.

che lei ha fatto nei confronti della nostra Guardia costiera, che ha lavorato bene, merita di essere considerata e lei lo ha fatto giustamente nel suo discorso. Sulla vicenda Diciotti, cari colleghi, hanno parlato tutti. Tutti si sono espressi. Molti sono stati riportati dai *media* nazionali ed internazionali, ma io vorrei cominciare il mio intervento con una riflessione che viene da una voce che non ha avuto, purtroppo, molta enfasi: la voce della comunità Eritrea in Italia. La comunità eritrea in Italia si è espressa con un comunicato stampa - datato, se non vado errato, 26 agosto - nel quale ha detto chiaramente che era molto dispiaciuta per quello che stava accadendo a bordo della nave italiana, ma era soprattutto dispiaciuta perché stava assistendo alla consueta strumentalizzazione politica delle persone ospitate su quella nave.

avevano preferito dare voce a coloro che vogliono tenere aperti i porti per aumentare i numeri dell'esodo dell'immigrazione clandestina. La stessa comunità eritrea ricordava che - spesso e volentieri - hanno provato a lottare strenuamente - e si impegnavano a continuare a farlo affinché in Italia i loro concittadini potessero entrare per vie legali, ove è consentito dal diritto internazionale, e a fare di tutto perché venissero fermate le morti in mare.

È un obiettivo che ritengo tutti i Gruppi politici condividano, così come lo condivide ogni cittadino italiano. Ma per non avere più un caso Diciotti bisogna necessariamente sviluppare le conseguenze che tale affermazione comporta. Non avere più un caso Diciotti dal mio punto di vista significa fermare il traffico di esseri umani: fermare il traffico di persone che non significa fermare le persone. Non avere mai più un caso Diciotti significa fermare l'immigrazione illegale, non i migranti. Ma come possiamo arrivare a questo?

che possa porre le basi di un progetto per la creazione di un nuovo Stato libico. Il nuovo Stato libico è l'unica strada che permette di stroncare il *racket* gestito dalle milizie. Stroncare il *racket* gestito dalle milizie significa anche ricostruire forze armate libiche unitarie; significa anche potenziare il lavoro della Guardia costiera libica, e su questo almeno il Senato e la Camera dei Deputati hanno dato un contributo con l'approvazione dell'utilizzo di nostre imbarcazioni a sostegno della Guardia costiera. Soprattutto significa rendere finalmente la costa libica un porto sicuro, in maniera tale che si possa bloccare fin dall'inizio la partenza in osservanza delle convenzioni internazionali.

«TV del dolore», sperimentato per la prima volta in Italia durante la tragedia di Vermicino, quando il piccolo Alfredino Rampi morì nel pozzo. Da quel momento in poi i *media* italiani si sono lasciati andare a una descrizione del dolore, spesso e volentieri a mio modo di vedere,

Un autorevole quotidiano nazionale ha riportato la testimonianza di una di queste persone, che dichiara essere arrivato su un barcone a seguito del pagamento di circa 10.000 euro, ottenuti con la vendita della casa materna e con il contributo degli zii che vivono in Svizzera. Dice questa persona di sentirsi in debito nei confronti dei suoi zii, che hanno contribuito con il pagamento ad un noto trafficante eritreo di 2.000 euro, in prima battuta, e poi di altri 8.000. Nell'articolo del quotidiano italiano si utilizza questa narrazione per far leva ancora sul meccanismo del dolore, che serve a trasfigurare la realtà. Quello che il Governo italiano sta facendo e che tutti i Governi dell'Unione europea dovrebbero fare è trovare un meccanismo automatico, consolidato ed efficace per impedire che questi criminali, i trafficanti di esseri umani che hanno base in Libia, in Eritrea e in altri Paesi del continente africano, possano permettersi di sfruttare la disperazione delle persone. Sono d'accordo con quanto diceva il Presidente del Consiglio: l'obiettivo è proprio quello e si può raggiungere soltanto con una concertazione internazionale e la concomitante

Etiopia ed Eritrea. E sono altre le condizioni che potranno permettere al nostro Governo di operare in maniera efficace e di provare a imporre all'Unione europea, che deve procedere deve procedere in maniera concorde con gli interessi dei Paesi che la compongono, di bloccare le emergenze migratorie. Ritengo non sia utile una militarizzazione dei confini europei, così come proposto da un autorevole esponente del Governo tedesco nelle scorse settimane e poi ripreso da Juncker. Ritengo piuttosto che occorra lavorare in maniera condivisa per un ricollocamento automatico ed obbligatorio delle persone che chiedono giustamente - perché ne hanno diritto - l'asilo in Europa: automatico e obbligatorio significa che devono accettarlo tutti i Paesi dell'Unione europea,

necessariamente parlare con tutti gli attori coinvolti, considerando i rischi che questo comporta; in secondo luogo, occorre provare a procedere alla trasformazione delle milizie armate

voglio ricordare che la Libia ad oggi non ha ancora sottoscritto la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati. Senza la sottoscrizione di quella Convenzione da parte del Governo libico nei prossimi mesi, nei prossimi mesi, diventa praticamente impossibile che il riconoscimento dello *status* di rifugiato venga effettuato direttamente nel Paese da cui si originano i flussi e poi attribuito al Paese che deve ospitarli. I Paesi devono accogliere questi flussi, quando sono legittimamente necessari e previsti dalle convenzioni internazionali, ma dobbiamo fare in modo che i Paesi di partenza abbiano gli strumenti per poterlo fare.

che l'atteggiamento della Presidenza nei confronti di questo Gruppo è assolutamente inaccettabile, includendo la sua interpretazione o la sua invenzione di articoli del Regolamento che non esistono. Io solleverò tale questione di fronte al Consiglio di Presidenza. Non possiamo prendere lezioni da chi ha occupato i banchi del

Ho chiesto a che titolo sta parlando e non lo ha ancora detto. La ringrazio,

io? Mi sembra che il compito della Presidenza sia quello di prevenire disturbi e assicurare che ciascuno possa parlare.

non la vuole? Non c'è stata alcuna invenzione. Le ricordo che l'articolo 85, sul posto degli oratori, così recita: «Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi». Questo articolo è stato sempre interpretato nel senso

finestra") sulla prevista nuova normativa relativa ai certificati di efficienza energetica. il meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi, come gli altri strumenti di promozione dell'efficienza energetica, è volto a stimolare interventi virtuosi di risparmio energetico nonché di effìcientamento dei processi produttivi e delle infrastrutture. Ciò rappresenta un vantaggio per tutto il sistema Paese, ivi compresa l'intera platea dei consumatori. Infatti l'efficienza energetica contribuisce contemporaneamente al raggiungimento degli obiettivi di: riduzione dei costi energetici, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della sicurezza energetica oltre a costituire un fattore di grande stimolo della crescita sostenibile. Il meccanismo dei certificati bianchi è disciplinato da decreti interministeriali MISE-MATTM, i quali fissano periodicamente per i distributori di energia elettrica e gas gli obiettivi nazionali di efficienza da raggiungere, nonché le modalità di riconoscimento dei certificati stessi corrispondenti al risparmio prodotto, che vengono commercializzati attraverso una piattaforma di scambio gestita dal Gestore dei mercati energetici (GME). L'ultimo decreto di definizione degli obiettivi e delle modalità è dell'11 gennaio 2017. Sul punto si osserva che tale meccanismo aveva dato chiari segnali di difficoltà nella capacità di raggiungere gli obiettivi di efficienza prefissati e aveva registrato fortissimi aumenti di prezzo, senza vantaggi per la politica dell'efficienza energetica e con un impatto negativo sui prezzi dell'energia elettrica e gas. I maggiori oneri sostenuti dai distributori per l'acquisto dei certificati sono stati altresì riconosciuti dall'Autorità per l'energia. In particolare, la capacità di generazione annua di certificati bianchi ha subìto una progressiva riduzione rispetto alle previsioni elaborate alle previsioni elaborate al momento della definizione degli obiettivi, poi confluiti nel decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Su questo può aver avuto un'incidenza il ritardo nell'emanazione e nell'entrata in vigore del decreto 11 gennaio 2017. Sul tema hanno avuto effetto anche gli esiti di indagini della magistratura su casi di emissione indebita di certificati bianchi legati alle cosiddette schede standardizzate, che nel 2017 hanno portato all'annullamento dell'emissione di un volume cospicuo di certificati. L'incrementata attività di controllo da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) sugli interventi eseguiti tramite schede standardizzate ha rilevato diffuse inadempienze e ha determinato un incremento elevato di respingimento delle domande presentate negli ultimi mesi, con annullamenti in autotutela di approvazioni già rilasciate, a partire dalla fine di giugno 2017, con un effetto di ulteriore riduzione dei certificati emessi. In questo contesto, nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018 il prezzo degli scambi di certificati bianchi avvenuti sul mercato regolato è salito di circa il 130 da un prezzo medio ponderato di 206,67 euro della sessione del 6 giugno 2017 a 479 euro nella seconda sessione di febbraio 2018.

alla fine del mese di febbraio il contributo tariffario stimato per l'anno 2017 risultava pari a circa 312 euro a certificato bianco. Tale valore, che eccedeva di oltre 120 euro il contributo tariffario concesso per il 2016, era destinato a salire ulteriormente e in modo totalmente slegato da un eventuale aumento del costo di produzione del risparmio e dai valori su cui erano state effettuate a suo tempo le scelte di investimento. La volatilità eccessiva dei prezzi stava, peraltro, frenando investimenti in grado di generare nuovi risparmi; dunque, la fluttuazione del prezzo, proprio perché percepita come eccessiva, stava anche mostrandosi inefficace mostrandosi inefficace nel riportare il sistema in equilibrio. Questa situazione era stata segnalata più volte dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per l'energia, cui era stato chiesto di valutare l'andamento del mercato e comunque, nelle more, di dare attuazione ai decreti interministeriali che, nel riconoscere all'Autorità il compito di definire il rimborso tariffario a favore dei distributori, prevedevano che questo fosse fatto nell'ambito di un valore massimo di riconoscimento. La previsione di porre un tetto massimo, soprattutto in una fase di mercato perturbato, avrebbe avuto l'effetto di frenare la rincorsa dei prezzi, ferma restando la necessità anche di altri interventi. L'Autorità per l'energia ha fornito una valutazione sull'andamento del mercato che non rilevava fenomeni atipici, mentre ha ritenuto di non definire un vero tetto al riconoscimento tariffario, che sostanzialmente seguiva l'andamento del mercato. A fronte di nuovi e ingiustificati rincari, di concerto con il Ministero dell'ambiente, è stato ritenuto necessario un intervento finalizzato a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta di titoli e a raffreddare la spirale dei prezzi, anche attraverso una diversa frequenza delle sessioni di scambio. Il solo annuncio del decreto correttivo agli inizi dell'anno 2018, accompagnato dal confronto con gli operatori coinvolti sulle misure in elaborazione, ha contribuito a calmierare le fluttuazioni di mercato, garantendo un effetto positivo sul contenimento degli oneri sulle tariffe dell'energia. I valori medi di scambio sono scesi progressivamente da 479 euro (febbraio 2018) a 350 euro (marzo 2018), per arrivare a 253 euro (giugno 2018). Tale valore di scambio è stato poi confermato nella sessione del 17 luglio 2018, la prima successiva all'entrata in vigore del decreto. Il provvedimento, dopo il parere favorevole dell'ARERA (delibera dell'11 aprile 2018) e l'intesa della Conferenza unificata, è stato emanato in data 10 maggio 2018, è stato registrato dalla Corte dei conti il 22 giugno 2018 ed è entrato in vigore Le altre modifiche introdotte, soprattutto sul lato dell'offerta, saranno oggetto di un attento monitoraggio, in quanto hanno bisogno di tempi maggiori per esplicare gli effetti attesi. Quanto ricostruito risponde alla prima osservazione dell'interrogante, relativa alla mancanza dei motivi di urgenza per l'emanazione delle nuove disposizioni. Naturalmente il Governo mantiene un monitoraggio attivo sull'evoluzione del meccanismo e potrà sempre intervenire per apportare modifiche al sistema. Riguardo alla definizione del valore massimo di riconoscimento, evidenzio che lo stesso fosse necessario, tanto che sia il decreto del 2017, sia il precedente decreto lo prevedevano esplicitamente, dando mandato all'Autorità di attuarlo. Si sottolinea, inoltre, che tale valore si applica al sistema nella sua interezza e non esclusivamente ai grandi inquinatori. Riguardo ai temi criticati del nuovo decreto, ritengo più equilibrato fornire una visione complessiva dei temi trattati, che vanno a favore del rilancio del meccanismo secondo criteri di maggiore razionalità. Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate. un insieme di modifiche interviene su aspetti tecnici o metodologici in grado di promuovere l'offerta di nuovi risparmi e semplificare le istruttorie da parte del GSE. In particolare, il provvedimento prevede la modifica del concetto di addizionalità e di *baseline*, al fine di renderla coerente con quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica. Inoltre, prevede la valorizzazione, in taluni casi, dell'energia fossile risparmiata a seguito dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'ampliamento della cumulabilità alla detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature, pur prevedendo un limite volto a evitare il rischio di sovraincentivazione. Sempre al fine di promuovere l'offerta, è poi aggiornata ed arricchita la tabella contenente le tipologie di intervento ammissibili, con circa trenta nuovi interventi. Con il decreto sono inoltre state approvate otto schede per la presentazione di progetti standardizzati, tra cui alcuni dedicati all'illuminazione pubblica, alle misure comportamentali e alla mobilità sostenibile con particolare riferimento all'acquisto di flotte di veicoli ibridi ed elettrici. Si differenziano inoltre i valori di vita utile da concedere agli interventi di nuova installazione, rispetto a quelli di sostituzione. Altre modifiche riguardano le modalità di adempimento da parte dei soggetti obbligati, in particolare in termini di maggiore flessibilità temporale. Infine, ulteriori modifiche integrano la regolazione economica del mercato centralizzato dei certificati in modo più efficace rispetto alla situazione attuale e introducono misure minime di trasparenza sui soggetti che partecipano al mercato stesso. In particolare, è prevista l'introduzione di un valore massimo unitario di riconoscimento per il contributo tariffario concesso ai soggetti obbligati, pari a 250 euro. Tale valore è stato quantificato con riferimento all'entità media degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, richiesta di incentivazione ai sensi del meccanismo dei certificati bianchi. È stata anche prevista la possibilità di bilanciare, ma a costi calmierati per i consumatori, eventuali squilibri temporanei e parziali che dovessero verificarsi tra domanda e offerta di certificati tramite un'offerta integrativa da parte del GSE, che può quindi emettere a favore dei soggetti obbligati il numero di certificati bianchi necessari al fine di adempiere agli obblighi minimi annuali già a partire dal corrente anno d'obbligo. I soggetti obbligati possono riscattare tali somme entro un tempo determinato, a fronte della presentazione dei risparmi sottesi alla quantità di titoli emessi, per mezzo di certificati da essi generati. Ribadisco che il Ministero dello sviluppo economico, in stretta collaborazione con il Ministero dell'ambiente, continuerà

nell'ambito della nuova programmazione integrata in materia di energia e clima, che sarà sviluppata nei prossimi mesi e in cui il Governo definirà i *target* e gli strumenti al 2030 in materia di sostenibilità, competitività e sicurezza del sistema energetico.

quel decreto interministeriale, vista anche la situazione di un Governo che, di fatto, era in carica solo per gli affari correnti;

tecnicamente anche molto complessa potesse essere oggetto di una discussione anche, per esempio, nelle Commissioni competenti. Chiedo qui anche al presidente Girotto se mai sia stato

a dir poco perplessa, perché lei è venuto qui, a nome del Governo, a dire che il decreto interministeriale non solo non è stato fermato, ma avuto pieno corso anche con l'insediamento del nuovo Governo, fino alla pubblicazione anche in *Gazzetta Ufficiale*. I punti critici,

di fatto per favorire i grandi inquinatori e non incentiva certamente i soggetti virtuosi a effettuare investimenti in efficienza energetica. L'emissione dei

e incentivare gli investimenti in efficienza energetica. La stessa questione riguarda l'aumento a due anni del tempo massimo per adempiere agli obiettivi minimi di efficienza. Al di

la collocazione geografica del Corno d'Africa ha da sempre conferito a tale regione una notevole rilevanza strategica, accompagnata da una tradizionale instabilità. La situazione di "né guerra né pace" tra Etiopia ed Eritrea ha costituito per lunghi anni uno dei fattori di criticità, risultando un ostacolo alla stabilità politica ed allo sviluppo regionale. La recente nomina del nuovo *premier* etiope Abiy Ahmed, il più giovane *leader* africano, ha costituito un elemento di svolta. Abiy ha impresso una decisa spinta riformista, sia all'interno dell'Etiopia sia a livello regionale, volta tra l'altro ad una normalizzazione delle relazioni con l'Eritrea. A tal proposito, la decisione di applicare pienamente l'accordo di Algeri del 2000 e le disposizioni della commissione arbitrale per la demarcazione del confine con l'Eritrea ha fornito il primo determinante impulso verso la riconciliazione. A seguito di una missione ad Addis Abeba di una delegazione governativa eritrea di alto livello guidata dal consigliere politico del presidente Afewerki, Yemane Ghebreab, e dal ministro degli esteri Osman Saleh, il primo ministro Abiy si è recato in visita ad Asmara lo scorso 8 luglio. Durante la visita, nella quale si sono avute manifestazioni popolari di giubilo senza precedenti, i due *leader* africani hanno convenuto di ristabilire le relazioni diplomatiche e di inaugurare una fase di cooperazione a tutto campo. La visita di Abiy ad Asmara è stata ricambiata da quella del presidente eritreo Afewerki ad Addis Abeba. I due *leader* congiuntamente hanno ribadito l'impegno a stabilire un partenariato completo e mutualmente vantaggioso ed hanno presenziato alla storica cerimonia di riapertura dell'ambasciata eritrea ad Addis Abeba. Inoltre, proprio ieri, i due *leader* hanno preso parte alla cerimonia con la quale è stato riaperto il confine fra Etiopia ed Eritrea, chiuso da anni di guerre. Gli elementi costitutivi di questo inedito scenario sono racchiusi in una dichiarazione di pace e amicizia. Tale documento, firmato congiuntamente dai due *leader*, si basa su cinque punti programmatici: formalizzazione della fine del conflitto; promozione di una stretta cooperazione in ambito culturale, sociale, economico, politico e di sicurezza; ripresa dei rapporti diplomatici e ripristino del commercio, delle comunicazioni e dei collegamenti; rispetto dell'Accordo di Algeri sui confini; cooperazione in ambito regionale a favore della pace e dello sviluppo. Una Commissione mista, presieduta dai due Ministri degli esteri, è stata incaricata di attuare le disposizioni della predetta dichiarazione di pace. contenute nella dichiarazione segnerebbe una svolta storica nei rapporti tra Etiopia ed Eritrea, determinando l'uscita di quest'ultima dall'isolamento regionale degli ultimi anni e la conseguente crescita degli scambi commerciali, premessa fondamentale anche per l'avvio di dinamiche di sviluppo che potrebbero condurre, specie in Eritrea, alla diminuzione dei flussi migratori verso l'Europa. La positiva dinamica tra Addis Abeba e Asmara sta generando importanti conseguenze anche sul piano internazionale e regionale. Infatti, a suggellare la nuova fase dei rapporti tra Etiopia Eritrea, il primo ministro Abiy ha richiesto al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, in visita ad Addis Abeba lo scorso 9 luglio per un incontro con i vertici dell'Unione africana, di farsi anch'egli promotore della revoca delle sanzioni verso l'Eritrea. Parallelamente, la delegazione etiope, capovolgendo radicalmente la storica posizione di Addis Abeba di chiusura sul *dossier* sanzionatorio, ha promosso un'analoga iniziativa a New York, nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sarà chiamato a discutere formalmente la questione

tratta di un'accresciuta interlocuzione che ha condotto, in primo luogo, alla storica visita ad Asmara, alla fine dello scorso luglio, del presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed, primo Capo di Stato somalo a recarsi in Eritrea dall'indipendenza del Paese. La ripresa delle relazioni diplomatiche, suggellata anche dalla firma di una dichiarazione di amicizia, ha aperto una nuova fase nei rapporti tra Asmara e Mogadiscio. Tale positiva dinamica si è arricchita nei giorni scorsi a seguito della visita congiunta del *premier* Abiy e del Presidente somalo, entrambi in visita ad Asmara per colloqui con il capo di Stato Afewerki. Tale incontro ha condotto alla firma di un accordo tripartito che prevede l'avvio di una collaborazione in campo politico, economico, sociale e culturale, in quello della sicurezza, anche attraverso l'istituzione di una Commissione congiunta di alto livello per coordinare gli sforzi nel quadro degli obiettivi dell'accordo. È indubbio che tale processo, dagli esiti comunque non del tutto scontati, potrà generare molteplici benefici, in primo luogo avviando dinamiche di sviluppo economico che potrebbero incidere su tutta la regione e diminuire i flussi migratori in partenza. In secondo luogo, la collaborazione regionale nel settore della sicurezza potrebbe consentire un miglior coordinamento in Somalia nel contrasto al terrorismo di Al Shabaab e Daesh. Per l'Italia, il Corno d'Africa costituisce da sempre una fondamentale priorità strategica. I trascorsi storici dei legami con Etiopia ed Eritrea conferiscono alle relazioni tra l'Italia e i due Paesi una dimensione di alto profilo e di speciale amicizia che, nelle numerose occasioni di interlocuzione, è stata ampiamente riconosciuta dalle controparti. Giova ricordare che la prima visita del presidente Mattarella in Africa si è svolta proprio in Etiopia nel marzo 2016 e che abbiamo mantenuto attivi i canali di dialogo con l'Eritrea, malgrado l'isolamento del Paese. Come già sottolineato dal vice ministro Del Re al vice ministro etiopico Hirut Zemene nel corso dei colloqui bilaterali avvenuti a Bruxelles lo scorso luglio, l'Italia incoraggia e sostiene questo nuovo processo, da cui trarranno sicuramente beneficio i due popoli. Anzitutto, il nostro Paese riserva al processo di riconciliazione tra Etiopia ed Eritrea la più alta attenzione dal punto di vista politico e intende avallare e sostenere gli sviluppi in corso con una serie di iniziative concrete. A tal fine, il presidente del Consiglio Conte ha rivolto al *premier* Abiy un invito a venire in Italia in visita ufficiale anche per meglio individuare quegli ambiti in cui il nostro Paese potrà sostenere la normalizzazione In secondo luogo, è in programma un rafforzamento delle attività sostenute dalla cooperazione italiana nei due Paesi, individuando, insieme alle controparti etiopi ed eritree, quelle specifiche iniziative volte al consolidamento del processo di distensione in atto. Viviamo una fase storica senza precedenti per il Corno d'Africa, in cui possono prevalere assetti di pace e progresso socio-economico. Si tratta di un cammino complesso, cui 1'Italia è pronta a contribuire con iniziative in ambito europeo. A Bruxelles le iniziative del nostro Paese si sono sempre caratterizzate per promuovere una migliore comprensione dell'importanza di intervenire in Africa, e ancor più nel Corno d'Africa, per combattere le cause dell'instabilità - fragilità istituzionali, terrorismo, traffici illeciti, povertà - e favorire l'avvio di dinamiche di sviluppo. L'Italia, che tra i Paesi membri dell'Unione europea esercita nel Corno d'Africa un ruolo primario, non mancherà di intensificare i propri sforzi a favore della stabilità e dello sviluppo della Regione, nel solco di un radicato impegno che desideriamo estendere e intensificare.

dato che sediamo all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - in merito alle richieste del Governo etiope di eliminare le sanzioni nei confronti del Governo eritreo.

Perché non chiedete all'Unione europea di realizzare un Economic Partnership Agreement con il Corno d'Africa, dato che è l'unica area dell'Africa in cui non esiste ancora?

cosa intendete fare affinché le imprese italiane possano utilizzare al meglio il piano di investimenti esterno dell'Unione europea nei confronti dell'Africa, attivo nelle prossime settimane?

non basta descrivere la situazione, quando si parla di Corno d'Africa. Sono passati mesi e le cose accadono. Lì si sta combattendo anche una guerra geopolitica e geoeconomia, fortunatamente con l'arma della pace. Tutti noi sappiamo quanto la Cina sia aggressiva in Africa, soprattutto in Etiopia. A Gibuti è stato realizzato il porto cinese più importante, anche *offshore* militare, e l'azione di pace, credo sostenuta dagli Stati Uniti, serve anche a contrastare l'espansionismo cinese in quel territorio. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per un Governo che deve avere a cuore la Libia e il Corno d'Africa, come aree di prioritario interesse strategico del nostro Paese.

turismo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la tutela e la valorizzazione del patrimonio arboreo monumentale italiano rientrano tra le priorità che intendiamo perseguire. Si tratta di una ricchezza unica, contraddistinta dal forte legame tra identità e territori,

Molise, Piemonte e Sardegna) gli alberi monumentali riconosciuti in Italia sono 2.734. Gli esemplari che ne fanno parte si caratterizzano per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, *habitat* per alcune specie di animali), per l'importanza ambientale, storica e culturale che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio, sia in termini estetici che identitari.

propositiva della procedura e di salvaguardia degli esemplari meritevoli di tutela. Rilevo al riguardo che l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, oltre ad esplicitare la definizione di "albero monumentale", ha istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al fine di garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge ne vieta l'abbattimento e le modifiche dei relativi apparati; solo in circostanze motivate e improcrastinabili, previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio vincolante del Corpo forestale dello Stato, può essere consentito l'abbattimento. Ricordo che, in attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016, la competenza assegnata dalla legge n. 10 del 2013 al Corpo forestale dello Stato in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali è stata trasferita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al del decreto ministeriale del 23 ottobre 2014, al censimento degli alberi monumentali del territorio di competenza e alla trasmissione dei conseguenti esiti alle Regioni. Ad esse spetta redigere, dopo l'istruttoria di competenza, un elenco regionale di alberi monumentali da inserire, previa verifica formale, nell'elenco nazionale in questione. Ciò posto, riguardo alla specifica fattispecie evidenziata dall'interrogante, per quanto di competenza del MIPAAFT, rilevo che gli alberi siti nella zona di riqualificazione viaria nel Comune di Matera non risultano iscritti nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, né risulta che il Comune abbia presentato alla Regione Basilicata alcuna proposta di monumentalità per gli stessi esemplari, ai fini di un prossimo inserimento. Peraltro, da informazioni assunte dal Ministero per i beni e le attività culturali, è emerso che in sede di conferenza di servizi indetta il 7 settembre 2017 dal Comune di Matera per l'espletamento dell'*iter* autorizzativo del progetto, la la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, in accordo con il Comune di Matera, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, prescrivendo che le essenze di pino espiantate su via Lanera vengano sostituite con essenze arboree da definire in fase esecutiva con la stessa soprintendenza. La suddetta prescrizione è stata recepita con atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Matera - settore manutenzione urbana ufficio verde pubblico in data 24 aprile 2018, con il quale si dispone che le 86 essenze arboree da abbattere andranno sostituite con un numero totale di 430 alberature, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento di tutela del verde urbano, fatta salva la rideterminazione numerica di tali alberature a seguito della perizia integrativa e fermo restando il rapporto di uno a cinque tra gli abbattimenti e le ripiantumazioni, che dovrà essere comunque rispettato. Il reimpianto *in loco* delle prime 60 essenze arboree dovrà avvenire entro e non oltre l'autunno del 2018.

Signor Presidente, ringrazio il Governo per avere preso a cuore la vicenda, a dimostrazione della sensibilità che questo Governo mostra verso la tutela verso la tutela dell'ambiente. Non altrettanto si può dire circa i Comuni, uno tra tanti quello di Matera che dovrebbe dimostrare maggiore sensibilità per la cultura del verde, anche alla vigilia di questo importante appuntamento come capitale della cultura 2019. Abbiamo dovuto registrare che tutta la comunità si è dovuta coalizzare per impedire che un provvedimento così poco condiviso e così poco democratico per la città potesse pregiudicare l'abbattimento se non di piante monumentali, quantomeno dei pini marittimi situati in area sottoposta a vincolo paesaggistico. È di questi giorni la notizia di un ripensamento da parte del Comune di Matera, con una variante che è stata presentata a seguito dell'attività svolta dalle organizzazioni ambientaliste locali e dai comitati cittadini, per cui ci sarà un ridimensionamento dell'opera, che probabilmente porterà anche a una riduzione dell'abbattimento delle piante. L'impegno assunto dall'amministrazione è di curare in maniera selettiva e chirurgica l'asportazione solo delle piante un po' più compromesse, cercando di

Signor Presidente, onorevoli senatori, il 27 settembre 2018 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, possa contenere misure tali da non pregiudicare in alcun modo l'eccellenza dell'*export* agroalimentare italiano. Al riguardo, sebbene la questione coinvolga i profili di competenza di più Ministeri, è utile soffermami in via prioritaria sugli aspetti propri del Ministero della salute, i quali risultano indubbiamente centrali nel tema in esame. Preliminarmente, faccio presente che l'Italia, anche dal punto di vista sanitario, si prefigge, tra i suoi obiettivi principali, quello di porre in essere azioni decisive volte ad affrontare la rilevante questione della malnutrizione in eccesso, tenendo in ovvia considerazione le influenze su di esse delle politiche economiche nonché le disuguaglianze sociali. Posto che tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la realizzazione o il rafforzamento di strategie e programmi che promuovono stili di vita salutari e la prevenzione delle malattie croniche, con speciale enfasi verso i i determinanti di salute, nonché attraverso l'implementazione di strategie multisettoriali a livello nazionale e locale, l'Italia considera prioritario contrastare i fattori di rischio e promuovere i determinanti con effetti positivi, attraverso tutti i possibili investimenti in termini di prevenzione e in interventi multisettoriali, i quali coinvolgono più amministrazioni pubbliche e la stessa società civile. Al fine di garantire tali priorità, l'Italia ha, dunque, tutto l'interesse a svolgere un ruolo importante nel quadro internazionale. A conferma di ciò desidero far presente che, in occasione dell'High Level Meeting dedicato alla prevenzione e al contrasto delle malattie non trasmissibili, che si terrà a New York il 27 settembre, l'Italia svolgerà il ruolo di co-facilitatore insieme all'Uruguay per garantire il massimo supporto al Ministero degli esteri in questo ruolo strategico, il Ministero della salute ha istituito una apposita *task force* per gli affari ONU. Già dallo scorso aprile, il Ministero della salute si è espresso sul testo in negoziato, appoggiando le politiche intersettoriali volte a promuovere stili di vita salutari, attività fisica regolare e diete sane, equilibrate e sostenibili. In questo contesto è stata espressa una posizione contraria alla demonizzazione di specifiche categorie alimentari oltre che ad ipotesi di etichettature, di avvisi e immagini volte a segnalare un pericolo correlato a specifici alimenti. Sottolineo che per quanto riguarda le politiche fiscali in campo alimentare, la posizione italiana è orientata ad eliminare del tutto il riferimento nel testo del negoziato, o, qualora ciò non fosse possibile, ad attenuarne il significato attraverso l'uso di un *wording* che segnali la volontarietà della misura, nonché l'eventuale applicazione in conformità alle politiche nazionali. Conforta peraltro che tale posizione sia condivisa anche da molti altri importanti paesi quali Stati Uniti e Giappone. Devo far presente, comunque, che il negoziato per la definizione del testo è ancora in corso e, anche allo stato attuale, questo Ministero continua a fornire gli elementi di competenza per supportare la scelta degli *statement* più opportuni per promuovere gli stili di vita salutari. È opportuno segnalare che il Ministero della salute da sempre promuove, in ogni consesso internazionale, la dieta mediterranea caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca e verdura, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, per i suoi effetti positivi sulla salute, e incoraggia produttori a mantenere la qualità eccellente dei prodotti tradizionali italiani. In linea con i più consolidati orientamenti scientifici, infatti, si è sempre considerata fondamentale la totalità della dieta e non il singolo alimento, non essendo possibile classificare gli elementi in buoni e cattivi poiché devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una semplice valutazione standardizzata. A tal proposito si può affermare che la riduzione di particolari nutrienti, ad esempio zuccheri e grassi, attraverso l'individuazione di semplici *target* numerici, non può essere condivisa non solo perché di difficile realizzazione ma anche perché di dubbia efficacia. Ciò che bisogna combattere sono, infatti, le abitudini scorrette e non il singolo alimento. Il Ministero della salute vuole accompagnare la popolazione verso un'alimentazione rapportata al tipo di vita che si conduce, considerando anche una serie di fattori quali età, sesso, attività fisica svolte allo stesso tempo, educando alle giuste quantità e alla variabilità delle porzioni. Non vi è dubbio che vi sia una crescente tendenza ad utilizzare indicatori che non sempre hanno una base scientifica, demonizzando anche singoli ingredienti, come grassi e zuccheri, senza considerare che esistono tecniche di cottura che possono incidere sulla composizione degli elementi e modificarne la qualità nutrizionale. Proprio tale tendenza è quella che fa temere che possano essere penalizzati taluni alimenti che fanno parte della dieta mediterranea e che ormai sono apprezzati in tutto il mondo. L'orientamento del Ministero della salute, perciò, è quello di evitare sistemi di valutazione basata sui meri profili nutrizionali o su rappresentazioni grafiche

un tavolo di lavoro a cui partecipano diverse amministrazioni, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, il MISE stesso ed associazioni di categoria, finalizzato alla definizione di una posizione nazionale sulle espressioni sintetiche delle informazioni nutrizionali in grado di considerare le peculiarità dei prodotti nazionali e bilanciare le informazioni sugli elementi nutrizionali con un più ampio riferimento al contesto generale della dieta e dello stile di vita mediterraneo. Il tavolo ha anche ipotizzato una proposta di modello supplementare di etichettatura nutrizionale che si configura quale contributo ad offrire alla discussione comunitaria per assicurare un'applicazione corretta ed uniforme del regolamento UE 1169 del 2011. È particolarmente importante evidenziare che tale modello, rispetto agli altri sistemi già in atto, *Nutri-Score traffic light*, si differenzia poiché non individua la classificazione degli elementi sulla base della loro formulazione in termini di energia e nutrienti negativi e positivi e non induce il consumatore a scegliere scegliere quegli alimenti che, sulla base di una particolare classificazione, risultano avere il migliore impatto sulla salute. È utile inoltre aggiungere, con riguardo alle politiche fiscali, che sia il Ministero della salute che il MISE hanno avanzato forti perplessità sull'applicazione di eventuali tassazioni maggiorate, poiché tale approccio, privo di alcuna componente educativa verso sane abitudini alimentari, può determinare un possibile spostamento dei consumi verso prodotti più economici e di scarsa qualità qualità nutrizionale, in particolare nell'età infantile ed evolutiva. In conclusione, desidero assicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero della salute, nel condividere le preoccupazioni espresse con il presente atto ispettivo, è intervenuto tempestivamente, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, affinché il negoziato ancora in corso possa dare un rilievo primario agli interventi basati sugli stili di vita, evitando considerazioni che non sono supportate da una forte

concreto, direi la minaccia, che quel documento preparatorio rappresentava nei confronti di prodotti di punta del nostro *made in Italy* (il prosciutto di Parma, il parmigiano Reggiano,

allarme, a nostro avviso assolutamente ingiustificato, produca poi una contrazione drastica nelle vendite. Di qui l'allarme giustificato di imprese e di lavoratori italiani. Il Governo in questa sede ci ha detto che sta intervenendo con misure che ritengo

o di altri alimenti naturali. Credo che questa sia la strada giusta. Mi auguro che il Governo abbia predisposto, come ci ha detto in questa sede, tutte le contromisure necessarie a sventare tale minaccia nei confronti del settore che in questo momento sta trainando, per aumento

ma anche di enogastronomia italiana.